Voteranno per primi gli onorevoli senatori. Pertanto, la programmata seduta pomeridiana di sindacato ispettivo non avrà luogo.

Signor Presidente, colleghi, la mozione in esame trae origine - e intende fornire un fattivo contributo parlamentare - dal processo in corso di ripensamento della Politica agricola comune europea. Infatti, come tutti sappiamo, l'applicazione dell'attuale sistema degli aiuti diretti di cui al primo pilastro, di quelli indiretti a progetto del secondo pilastro e dell'organizzazione comune di mercato hanno evidenziato criticità in vari Paesi europei, tra cui l'Italia. Oggi ci troviamo nuovamente in una fase di consultazione, per comprendere quale direzione imprimere alla Politica agricola comune dal 2020 in poi, tenendo ben chiari alcuni punti fondamentali, che nel caso in questione - quello dell'agricoltura - sono assolutamente fondamentali per la stessa qualità della vita delle persone. Il primo punto che la politica agricola deve garantire è certamente quello della sicurezza alimentare. L'Unione europea ha 500 milioni di consumatori che richiedono tutti un regolare approvvigionamento di alimenti sani e nutrienti a prezzi accessibili. Ma in agricoltura non conta solo la quantità. La nuova PAC, quella che stiamo delineando, dovrà promuovere sempre più la qualità e la diversità, rispettando l'ampia varietà di tradizioni agricole dell'Europa, puntando in maniera più mirata al sostegno pubblico, riducendo il divario tra i pagamenti ai diversi Paesi e regioni dell'Unione europea e favorendo tutti i diversi tipi di aziende agricole e pratiche rurali. La seconda questione fondamentale che vogliamo tutelata dalla nuova PAC è quella del nostro ambiente e della biodiversità. Un uso attento delle risorse è essenziale per la produzione alimentare e per la nostra qualità di vita sia per il presente che per il futuro. Già oggi il 30 per cento dei pagamenti diretti è legato a pratiche sostenibili ed ecocompatibili, ma questa quota va, a nostro giudizio, aumentata. Il terzo fattore è la vitalità delle campagne. Vogliamo che la PAC sviluppi un'azione volta a preservare e a incrementare la qualità e la vitalità delle nostre campagne, anche perché vi vivono e lavorano quote importanti della nostra popolazione. L'agricoltura e l'industria agroalimentare oggi significano 46 milioni di posti di lavoro e il 6 per cento del PIL europeo. Con questa mozione, dunque, ho voluto enucleare in punti specifici - e ringrazio i colleghi che l'hanno firmata con me con me - aspetti e caratteristiche che, secondo l'Italia, la PAC dovrà assumere nel nuovo volto che i negoziati a livello europeo dovranno delineare. Siamo ben consapevoli che, nonostante le progressive riforme con indubbi risultati positivi, permangono problemi che questa fase di negoziazione può risolvere. Entro nello specifico e concludo il mio intervento. Per quanto concerne l'Italia, vi è una dinamica strutturale che tende a ripercorrere di anno in anno un sistema che vede minime variazioni dei sostegni ad una platea costante di beneficiari. Tale dinamica dovrebbe, a nostro avviso, essere corretta consentendo apporti mirati e soprattutto ispirati a un'ottica di incentivo e premialità rispetto a incrementi di produttività e avanzamenti tecnologici e di qualità e redditività delle coltivazioni. Il tessuto economico del comparto primario italiano vede ancora la preponderanza di piccole e medie imprese, per le quali i sistemi di sostegno europeo si rivelano di difficile accesso, soprattutto per quanto concerne la politica di sviluppo rurale, ma anche per il sostegno accoppiato. Urge pertanto un intervento redistributivo che può essere attuato con diverse modalità. Il regolamento cosiddetto *omnibus*, che sta esaminando il Parlamento europeo, è sicuramente di primaria importanza, ma un sostrato imprescindibile è quello della semplificazione delle procedure di accesso agli aiuti e della riduzione degli oneri burocratici. Inoltre, occorre vigilare affinché gli stanziamenti finanziari siano idonei a garantire l'attuazione di una politica prioritaria e fondamentale per l'intera Unione Nel contempo, ritengo che il nuovo sistema debba tutelare e garantire le peculiarità e le differenze delle agricolture europee, in seno alle quali quella italiana si caratterizza per produzioni di eccellenza e sovente di "nicchia", che sono la ricchezza del *made in Italy*. Anche la conformazione orografica e geologica del territorio nazionale pone in rilievo la necessità di identificare nuove modalità di gestione dei rischi ambientali. Ovviamente, colleghi, molti altri sono i temi toccati dalla mozione che ho inteso presentare. Auspico un'ampia condivisione da parte di tutti i colleghi dell'Assemblea. Il sostegno all'attività agricola costituisce infatti, a mio avviso, un tema trasversale rispetto al quale il Parlamento, con una posizione unitaria, può sostenere e orientare le scelte governative nazionali e quelle europee sovranazionali. Colleghi di tutti le forze politiche, non perdiamo l'occasione di dare un segno forte e unitario che sia anche di incoraggiamento per i nostri agricoltori. PRESIDENTE. Ha facoltà di

la Commissione europea e gli organi dell'Unione si trovano oggi ad affrontare un'ipotesi di riforma della riforma, a discutere di alcuni correttivi di rilievo ai testi regolamentari in vigore che avevano introdotto importanti innovazioni nell'impostazione e nella gestione degli aiuti, con l'obiettivo dichiarato di predisporre un maggiore orientamento al mercato delle aziende agricole. Questi correttivi evidentemente sono necessari, almeno in Italia, perché la PAC non ha finora portato ai risultati sperati, anche per alcune difficoltà specifiche del nostro Paese, prima tra tutte la cronica incapacità di spendere i fondi a disposizione. Nel cosiddetto nuovo regolamento *omnibus*, attualmente all'esame del Parlamento europeo, si prevedono tra l'altro importanti modifiche in materia di gestione dei rischi di mercato, la semplificazione delle procedure burocratiche, l'accesso agli aiuti per i giovani, la gestione del regime dei prodotti di qualità, la facoltà di disaccoppiare gli aiuti rispetto alla produzione in alcuni settori e di risarcire in modo più efficace i danni da calamità naturale. Non si possono non evidenziare, in questa sede, alcuni dei problemi non risolti dalla riforma della PAC e alcune problematiche ulteriori derivanti dall'applicazione concreta che è stata disposta per il nostro Paese. La PAC non ha ad oggi risolto adeguatamente i problemi di sperequazione nella distribuzione dei fondi a danno delle piccole aziende che pure costituiscono, tuttora, una rete territoriale insostituibile per la produzione del cibo e la tutela della biodiversità agraria. Nel nostro Paese le aziende agricole che ricevono fino a 5.000 euro all'anno sono l'87 per cento del totale e hanno incassato appena il 26 per cento dei fondi stanziati, mentre il restante 13 per cento delle aziende riceve i due terzi dell'aiuto pubblico. L'attuazione della riforma non ha arrestato il fenomeno di concentrazione oligopolistica delle aziende che forniscono le sementi, i macchinari e i mezzi tecnici per l'agricoltura e che controllano le piattaforme della grande distribuzione: fenomeno in preoccupante crescita che contribuisce alla perdita di potere negoziale e di reddito per gli agricoltori lungo le filiere e al costante ampliamento della forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo del prodotto. Infine, l'applicazione tecnica della riforma non ha prodotto, ad oggi, le attese semplificazioni burocratiche a favore degli operatori agricoli, che rimangono invece costantemente e fortemente soggetti a un sovraccarico di oneri amministrativi che grava moltissimo sui loro bilanci. Occorre sottolineare inoltre che anche l'azione delle Regioni e degli enti erogatori nazionali non è esente da problematiche. Per effetto di ritardi organizzativi e di mancati controlli, la Commissione europea si appresta - ad esempio - a imputare all'Italia, negandone la liquidazione, parte dei fondi per lo sviluppo rurale assegnati per il periodo 2007-2013, per un totale di un miliardo e 700 milioni di euro. Dai dati diffusi recentemente dalla Commissione europea, si evince inoltre che l'Italia, con il 6,2 per cento dei fondi erogati ai beneficiari al 31 dicembre 2016, si colloca al penultimo posto all'interno dell'Unione europea per la quota di risorse comunitarie spese per gli interventi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con un preoccupante ritardo nella capacità di spesa che non arriva nemmeno alla metà della media europea, pari al 14,2 per cento. Nel dispositivo della mozione a mia prima firma si propongono una serie di indirizzi per orientare l'azione del Governo nella trattativa in corso sui correttivi da apportare alla riforma della PAC. in primo luogo ribadire, in sede europea, la rilevanza strategica della PAC quale strumento finalizzato a garantire l'approvvigionamento alimentare europeo e assicurare l'invarianza delle risorse già assegnate agli Stati membri. Chiediamo al Governo di intervenire sull'orientamento degli aiuti al fine di assicurare un supporto adeguato alle aziende contadine a conduzione familiare e prevedere misure finalizzate al contrasto dei fenomeni di eccessiva concentrazione e di oligopolio nella fornitura delle

senso. Ha facoltà di parlare il senatore Candiani per illustrare la mozione n. 761.

di impegnare il Governo ad approfittare dell'occasione del regolamento *omnibus* di aggiornamento della PAC attuale per concentrarsi soprattutto sulla PAC *post* 2020 e, in particolare, a convogliare gli sforzi sulla stabilizzazione dei mercati, sul funzionamento della filiera alimentare, sulla salute degli alimenti e sull'occupazione. Chiediamo un impegno al Governo affinché il regolamento *omnibus* e, soprattutto, la riforma PAC *post* 2020 siano l'occasione per realizzare una vera e propria semplificazione della vita dei nostri agricoltori, parte attiva della Politica agricola comune. Chiediamo ancora che il Governo si impegni a rendere disponibili le statistiche ufficiali sul numero dei beneficiari, sulla distribuzione delle risorse, sui valori dei pagamenti, sulle superfici e sui capi ammissibili, necessarie a svolgere analisi e ragionamenti per poi procedere, a ragion veduta, a una revisione di un'impalcatura normativa che può e deve essere migliorata nell'interesse dell'agricoltura italiana. Chiediamo altresì al Governo che si impegni a precisare, durante l'esame delle modifiche correttive da apportare al regolamento sullo sviluppo rurale, che, per quanto riguarda la fissazione delle soglie per l'accesso ai premi per il primo insediamento dei giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, questa sia facoltativa per gli Stati membri che ogni anno provvedono a notificare le modifiche,

precluso l'accesso alla misura a un notevole numero di aziende che pure avrebbero avuto diritto a ricevere il sostegno. Chiediamo poi al Governo di prendere impegno affinché sia previsto che il contributo dello sviluppo rurale per finanziare gli strumenti di stabilizzazione del reddito non solo riguardi gli indennizzi pagati

unicamente nella misura necessaria ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione, nonché prevedere che gli Stati membri possano modificare le precedenti scelte in materia di pagamento accoppiato,

Commissione europea affinché siano previste, nell'ambito dei pagamenti diretti, misure che tengano conto del valore aggiunto che le aziende, site nelle aree rurali dove il rischio abbandono è molto alto e dove l'agricoltura rappresenta un'importante fonte di reddito per la popolazione locale, forniscono all'economia del Paese; 8) a valutare strumenti di sostegno *ad hoc*, in termini sia di supporto economico che soprattutto di semplificazioni burocratiche, per favorire l'insediamento di nuovi e giovani agricoltori;

efficacia; 10) a far sì che sul secondo pilastro venga mantenuta la possibilità di erogare finanziamenti a fondo perduto sugli investimenti in azienda, come attualmente previsto, e non vengano trasformati questi interventi, limitandoli agli strumenti finanziari, poco efficaci e richiesti; 11) ad attivarsi, affinché chiediamo al Governo di attivarsi, affinché le norme, sia comunitarie che nazionali, siano stilate in modo semplice e chiaro, al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore semplificazione e alleggerimento burocratico delle procedure di attuazione della PAC. Questi sono gli impegni per i quali chiediamo al Governo di attivarsi nei confronti dell'Unione europea.

sul fatto che tutti dobbiamo convergere per aiutare a sviluppare una migliore politica agricola nel nostro Paese. L'agricoltura è sempre stata al centro della nostra attenzione. Non possiamo, però, non rilevare che da parte del Governo italiano occorrerebbe non solo

la cosiddetta Politica agricola comunitaria, riversata sui territori nazionali - in questo caso sul nostro Paese - abbia dinamiche assolutamente più efficaci. Mi riferisco, naturalmente, al ruolo del Governo di tramite dei fondi comunitari. Molto spesso questo tramite si rileva lungo, con una burocrazia eccessiva. Potrei fare l'esempio della Regione siciliana, dove ancora si attende che le contribuzioni relative al biologico del 2015 vengano erogate: neanche la prima annualità, infatti, è stata erogata. Quindi, signor Vice Ministro, sull'attività delle Regioni per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi comunitari. Non possiamo soltanto rimetterci alle norme, ma dobbiamo anche far sì che le norme, i provvedimenti e i regolamenti vengano attuati. una maggiore attenzione da parte del Governo sull'agricoltura italiana, che ha le sue specificità. E la nostra mozione individua tutta una serie di strumenti e di elementi essenziali che devono essere applicati all'agricoltura italiana. Mancando essi in un regolamento comunitario, dove naturalmente si guarda guarda di più ai massimi sistemi, ogni Paese dovrebbe compensare e completare con una attività nel suo territorio. In particolare ciò vale che non riceve i contributi dell'agricoltura professionale erogati dalla Comunità europea, e che è completamente abbandonata mentre è assolutamente importante per mantenere gli equilibri e gli assetti idrogeologici e ambientali. Nel nostro Paese la montagna è trascurata. Molto spesso la montagna è oggetto di agricoltura non professionale ma complementare rispetto anche ad altre attività lavorative. Ma è proprio quell'agricoltura che viene fatta con sacrificio dai non professionali che mantiene l'ambiente e gli assetti idrogeologici e dovrebbe essere oggetto dell'attenzione di una politica nazionale a completamento dell'attenzione che la politica comunitaria dedica ai grandi e medi imprenditori e, comunque, all'agricoltura cosiddetta professionale.

accusiamo una disattenzione del Governo su alcune specificità dell'agricoltura nazionale. Mi riferisco - ad esempio - ad alcuni trattati internazionali, condotti direttamente dal Governo, che consentono forti immissioni di prodotti extracomunitari sul mercato nazionale e, quindi, vanificano in parte lo stesso effetto regolatorio della Politica agricola comune per quanto riguarda, Abbiamo visto arrivare olio e agrumi per effetto di politiche del Governo italiano e non riferite alla

chiediamo con la nostra mozione, che è assolutamente in linea con l'interesse dell'Italia a mantenere una Politica agricola comunitaria efficace ed efficiente, ma che intende anche richiamare l'attenzione del Governo italiano sulle specificità della nostra agricoltura, che non sono le stesse dell'agricoltura continentale

giunge a metà del percorso: è, per così dire, a una sorta di giro di boa ed è condivisa da tutti l'esigenza di una sua revisione, che sia rivolta soprattutto a sanare alcune criticità evidenti per renderla più incisiva ed efficace. Questa fase di revisione di medio termine, peraltro, si innesta in un momento particolarmente delicato nella vita dell'Unione europea: la Brexit è attualmente un fatto che deve ancora declinare i propri effetti nei più diversi ambiti ma, per quanto riguarda il bilancio del settore agricolo dell'Unione, già sappiamo che ci costerà circa tre miliardi di euro all'anno. queste cifre sono accompagnate da echi sempre più forti rispetto a una possibile reintroduzione dei dazi provenienti da Oltreoceano. È bene ricordare, da questo punto di vista, come l'agricoltura sia uno dei collanti dell'Europa, innanzitutto per l'importanza che essa riveste negli impegni di bilancio europeo, costituendo quasi il 40 Per evidenti motivi di tempo, non procedo alla lettura della mozione, ma provo a illustrare quelli che ritengo gli impegni che mi auguro che il Governo condivida, promuovendoli in sede europea nel redigendo regolamento *omnibus*. Mi limito pertanto a riferire che le richieste contenute nella mozione sono riassumibili secondo due macrodirettrici: la semplificazione della macchina burocratica e, dall'altra, un più forte e irrobustito sostegno a chi fa agricoltura. Riguardo alla semplificazione della macchina burocratica, una nota particolare rileva e merita il *greening* che, senza timore di essere smentito, posso dire che scontenta tutti, essendo per lo più un aggravio per gli agricoltori in ragione dei vincoli e dei bizantinismi procedurali insostenibili che vanno assolutamente semplificati, senza produrre peraltro particolari effetti da un punto di vista della compatibilità ambientale. Nella mozione si chiede al Governo di prevedere una semplificazione delle sue regole e delle soglie fisiche attualmente previste, nonché una rivalutazione del beneficio ambientale che le pratiche collegate all'attuale *greening* possono garantire per il sistema agricolo e ambientale dell'Unione. Riguardo invece al sostegno a chi fa agricoltura, nella mozione si chiedono forme di tutela per così dire a ombrello: si va dalla richiesta di maggiore sostegno alla figura dell'agricoltore attivo a una maggiore implementazione degli strumenti di gestione dei rischi al fine di contribuire alla stabilizzazione dei redditi degli agricoltori, perché è un dato incontrovertibile che sono aumentati gli scenari dei rischi, dalla volatilità dei prezzi agli eventi climatici. Dobbiamo quindi dotare la PAC di un sistema di tutela e garanzia attualizzato; una tutela che deve essere declinata anche nei confronti della posizione di *price taker* che spetta all'agricoltore, troppo spesso schiacciato dalla grande distribuzione e dalla concorrenza sleale. Occorre quindi promuovere la valorizzazione del mercato dei prodotti agricoli attraverso certificazioni etiche e il rafforzamento di politiche contro le diverse forme di sfruttamento. Quanto brevemente riassunto e illustrato è espressione di indirizzi politici che convergono verso una sensibilità che ancora deve trovare modo di esprimersi compiutamente nella PAC. Faccio riferimento alla necessità che dovrà accompagnare e caratterizzare anche la futura programmazione, che si riassume nella sinergia da centrare e far crescere tra le politiche ambientali, la cui attuazione è delegata agli agricoltori, e le politiche di sostegno alla competitività aziendale dei sistemi agroalimentari. Concludo richiamando la necessità di far sì che gli agricoltori possano continuare a svolgere bene, anzi sempre meglio, la loro preziosa e insostituibile funzione di gestione delle terre, che rimane obiettivo fondamentale soprattutto in quelle aree geografiche più marginali, dove è l'agricoltura, attraverso i servizi ambientali e il sostegno economico, a rappresentare spesso l'unico, ma il più efficace freno allo spopolamento e al conseguente dissesto idrogeologico.

l'instaurazione di un mercato comune dell'Unione europea, finalizzato all'attuazione delle libertà relative alla circolazione di beni, servizi, persone e capitali è stata accompagnata e sostenuta, sin dall'avvio della Comunità europea, dall'introduzione di politiche comuni; la prima ad essere attuata e finanziata è stata proprio la politica agricola comune (PAC), da cui non si può prescindere per il rilancio della agricoltura italiana; con un bilancio annuo di circa 59 miliardi di euro, pari al 38 per cento del bilancio dell'Unione, la PAC rafforza la competitività e la sostenibilità dell'agricoltura della UE, finanziando una serie di misure di sostegno attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). In questo senso la competitività dell'Europa si gioca, in primo luogo, sul piano dell'innovazione e della coesione sociale. A tal fine il processo di revisione della PAC costituisce un'occasione importante per aprire la strada a strumenti più incentivanti e premianti a favore di chi si dedica effettivamente all'agricoltura, riducendo drasticamente i casi di rendita e adottando metodologie innovative e sostenibili. Detto questo, nel rivedere la PAC è soprattutto necessario renderla sempre più uno strumento di intervento preventivo a tutela degli agricoltori contro il doppio rischio rappresentato dall'instabilità dei mercati e dai cambiamenti climatici, restituendo ai produttori la necessaria autonomia operativa. Inoltre la politica di libero scambio, finora intrapresa dall'Unione europea, ha finito spesso per essere afflittiva per il comparto agroalimentare e discriminante per i prodotti europei. In realtà, le decisioni comunitarie dovrebbero essere assunte invertendo questo paradigma, e cioè attraverso un regime dei prezzi e un'attività normativa e di sostegno economico che valorizzino le produzioni europee e dei singoli Stati membri. Sul punto proprio i piccoli produttori agricoli e i piccoli trasformatori vivono una situazione assai difficile, spesso schiacciati tra la tirannia della grande distribuzione - da un lato - e l'indifferenza delle istituzioni - dall'altro e solo grazie al rapporto diretto con i consumatori, con gruppi di acquisto e mercati di filiera corta, riescono a trovare uno sbocco allo stato di crisi; una crisi che purtroppo è dovuta anche all'assenza di un concreto sostegno pubblico a favore dell'agricoltura familiare e delle lavorazioni degli artigiani del cibo di qualità. Proprio per questo sarebbe opportuno porre in essere appositi strumenti normativi e finanziari a favore dei piccoli produttori agricoli, che giorno dopo giorno rischiano di perdere i propri beni aziendali nell'ambito di procedure esecutive, comprese quelle legate alla costruzione di opere infrastrutturali. A tal proposito l'esempio della costruzione della TAP, in Puglia, rappresenta bene l'emblema dell'intera situazione. È inoltre opportuno prevedere un sistema di aiuti maggiormente vincolato all'apporto di lavoro garantito e al valore aggiunto prodotto in agricoltura, sempre al fine di rafforzare l'obiettivo finale della sostenibilità economica delle imprese, che si può costruire soltanto partendo dall'analisi effettiva della realtà in cui gli imprenditori operano. A ciò si aggiungono la necessaria sburocratizzazione delle procedure, la trasparenza nell'assegnazione delle risorse e la possibilità di verificarne la corretta destinazione oltre che l'utilizzo. In aggiunta, per la programmazione PAC *post* 2020, vanno ripensate le due componenti del *greening* e dell'aiuto accoppiato, al fine di procedere a una riallocazione delle risorse che consenta una maggiore efficacia delle misure stesse. Parte di tali risorse, infatti, potrebbe essere destinata a un fondo dedicato a finanziare interventi in caso di gravi squilibri di mercato a seguito di emergenze dovute a epizoozie, fitopatie (come la xylella fastidiosa, la botrite e il punteruolo rosso) calamità naturali e a erogare contributi finalizzati al rilancio di settori strategici in difficoltà, come quello olivicolo, cerealicolo e zootecnico. Concludendo, un un ruolo importante è rivestito dalla tracciabilità dei cibi, una tematica intorno alla quale ruotano altri importantissimi argomenti cruciali, quali l'obbligatorietà delle indicazioni dell'origine in etichetta, ma anche il tema delle filiere corte, del cibo locale e di stagionalità delle colture, aventi valore ambientale e paesaggistico. Si tratta di questioni che non possono essere tralasciate. La politica agricola, infatti, è anche e soprattutto politica alimentare. Per quanto si possa inseguire il profitto, l'uomo non può nutrirsi di banconote e solo orientando la politica agricola a una concreta sostenibilità e qualità la si potrà effettivamente proteggere

la politica agricola comune (PAC) è una delle politiche comunitarie di maggiore importanza, dal momento che impegna circa il 34 per cento del bilancio dell'Unione europea gli organi dell'Unione hanno radicalmente cambiato la politica tradizionale e, mentre in precedenza il reddito degli agricoltori comunitari veniva sostenuto principalmente a mezzo di sussidi, dagli anni '90 si è cominciato a dare maggiore applicazione al sistema delle "quote" di produzione, in modo da garantire agli agricoltori un livello minimo dei prezzi dei prodotti e di ripartire equamente tra i vari Paesi comunitari una quota di produzione garantita. Tale politica ha però avuto un esito sostanzialmente negativo, in particolare per l'Italia

per difendere le loro esigenze specifiche nel settore agricolo, a differenza di quelli dell'Europa settentrionale e della Francia, che hanno saputo volgere la Politica agricola comunitaria a proprio favore attraverso un'azione più incisiva e presente. Il primo pilastro della PAC è costituito dai pagamenti diretti, che si articolano in sette componenti, alcune delle quali devono essere attivate obbligatoriamente - come sappiamo - mentre altre hanno un regime facoltativo, in quanto rimane a discrezione degli Stati membri se attivarle o no, il tutto entro percentuali del massimale nazionale. Nella mozione presentata dal mio Gruppo, abbiamo affrontato vari temi: un comparto agricolo in grado di garantire un vero reddito agli agricoltori; una nuova valorizzazione delle aree rurali; di produrre alimenti garantendo la sicurezza alimentare e l'alta qualità legata al territorio e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio anche attraverso la promozione dell'uso di energia da fonte rinnovabile;

nonostante l'evoluzione della PAC (apprezzabile certamente il fatto che per il frumento duro ci sarà un aumento delle risorse per 8 milioni di euro e il pagamento passa da 67 a 75 euro

azioni facoltative (per esempio pagamento redistributivo per i primi ettari, pagamento delle aree svantaggiate eccetera) previste nel primo pilastro della PAC, le quali potrebbero rivelarsi degli straordinari strumenti per fronteggiare la crisi ciclica che attanaglia il settore promuovendo meccanismi di gestione amministrativa snelli, rapidi, chiari, intellegibili per tutti gli operatori, il più possibile sburocratizzati, consentendo così agli operatori non solo la profonda conoscenza delle possibilità della riforma, ma anche la facilità di accesso alle misure di sostegno;

il giovane imprenditore non può accedere, soprattutto per il muro che trova nel nostro sistema bancario. Bisognerebbe,

Governo a consentire che la politica comune europea giunga a riguardare tutte le fasi della filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione, intervenendo anche sull'organizzazione comune di mercato, favorendo e sollecitando idonee idonee misure di sostegno delle zone svantaggiate, mediante specifici strumenti, anche finanziari, per compensare le difficoltà strutturali e competitive che caratterizzano tali zone, anche alla luce dell'attuale assetto della ripartizione dei premi del primo pilastro della PAC, che non privilegia detti territori .

Presidente, onorevoli colleghi, la Politica agricola comune è uno dei progetti che devono rendere il nostro Paese fiero per aver contribuito a fondare l'Europa unita. Si tratta di uno di quei macro capitoli alla base della costruzione europea nel tempo, si è evoluto per andare incontro alle esigenze continuamente mutevoli della società, del sistema economico e, in particolare, del settore agricolo. Ci troviamo in un periodo storico che rappresenta un momento chiave per l'agricoltura europea, nel quale siamo chiamati a dare seguito alle esperienze più virtuose degli ultimi anni, a fare tesoro delle iniziative che hanno mostrato risultati meno positivi e a incoraggiare lo sviluppo imprenditoriale verso soluzioni innovative e tecnologiche. Come ricordato anche dalla mozione n. 744, presentata dal senatore Formigoni, vorrei fare riferimento alla proposta, avanzata nel settembre 2016 dalla Commissione europea, di un nuovo regolamento, cosiddetto *omnibus*, all'interno del quale è previsto un processo di revisione intermedio della PAC. In questo quadro, è stata lanciata a livello europeo una consultazione rivolta a cittadini, imprenditori e istituzioni proprio sul futuro della PAC: tutti sono chiamati a esprimersi sui profili di interesse dell'agricoltura europea, sui suoi lati positivi e su quelli più critici. In particolare, la nuova proposta legislativa della Commissione, che riassumerà i risultati della consultazione, perseguirà gli obiettivi della semplificazione e dell'alleggerimento degli oneri amministrativi nel comparto agricolo, dell'incentivazione dello sviluppo rurale, dei miglioramenti nell'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli. Come già detto tale regolamento *omnibus* non rappresenta una completa revisione della PAC, che attualmente si trova in una fase di transizione tra gli impegni assunti negli scorsi anni e quelli da assumere, in via riformatrice in futuro. Il provvedimento mira a introdurre alcune modifiche che riguardano proprio la semplificazione nei pagamenti diretti, la definizione di agricoltore attivo, il sostegno accoppiato facoltativo e il regime di pagamento unico per superficie e i giovani agricoltori. Mi vorrei soffermare proprio su quest'ultimo tema. Come ricorda anche la mozione presentata dal senatore Formigoni, gli obiettivi che dovranno essere perseguiti con il nuovo regolamento per investire nel capitale umano agricolo rappresentato dai nuovi agricoltori sono necessariamente quelli della diminuzione delle rigidità relativamente al credito e alla burocrazia, della estensione della definizione di giovane agricoltore e dell'attuazione di misure di sostegno alle imprese giovanili, che molto spesso sono quelle più innovative e investono maggiormente in ricerca e sviluppo e nuove tecnologie. La questione riguarda assai da vicino il nostro Paese. L'Italia è infatti il Paese europeo con il maggior numero di aziende agricole guidate da *under* 35, numero che supera le 50.000 unità. Nonostante ciò, tali imprese rappresentano solo una minima percentuale di quelle attive nel comparto agricolo e gli ostacoli alle aspirazioni dei tanti giovani che vogliono lavorare in agricoltura sono ancora numerosi: eccessiva burocrazia, difficoltà nell'accesso al credito e, soprattutto, scarsa disponibilità dei terreni. Secondo un'indagine di Coldiretti, la metà delle imprese agricole condotte da giovani ha bisogno di terra, in affitto o acquisizione, il cui costo medio è di circa 20.000 euro, un valore superiore a quelli di Germania e Francia. La media, tuttavia, è il risultato di forti asimmetrie presenti sul territorio nazionale, con valori che oscillano tra i 1.000 euro all'ettaro dei pascoli nella Provincia di Catanzaro e il milione di euro per un ettaro di frutteto o vigneto nelle zone di produzione più celebri, dalla Toscana al Trentino. In questo senso, sono estremamente positive due recenti iniziative istituzionali. La prima è dell'Agenzia del demanio che, nell'ambito dell'iniziativa Terrevive, ha deciso di mettere sul mercato, in vendita o in affitto, 630 ettari di terreni a vocazione agricola. In questo modo, con la collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si possono riportare a nuova vita i terreni a vocazione agricola e trasformarli in un'occasione di lavoro soprattutto per le nuove generazioni, dato che le aree sono messe a bando a prezzi calmierati e la normativa dedicata permette agli *under* 40 di avere diritto di prelazione. a oggi l'Agenzia ha individuato circa 1.500 terreni adatti a essere utilizzati per l'agricoltura o l'allevamento e ne ha già messi a bando quasi il 50 per cento, per un valore pari a tre milioni di euro. La seconda iniziativa riguarda la Banca delle terre agricole, prevista dal cosiddetto collegato agricolo, che si prefigge, attraverso una dettagliata mappatura, di favorire l'incontro tra domanda e offerta dei terreni e delle aziende agricole di natura pubblica. Sul sito dell'ISMEA, ente economico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, terreni e aziende in vendita sono descritti minuziosamente, a partire dai primi 8.000 ettari di terreni di proprietà dell'ISMEA stessa, e messi in vendita con una corsia preferenziale per i giovani. Mi fa piacere ricordare che il bando 2017 per il primo approccio di giovani in agricoltura che intendono acquistare un'azienda agricola prevede mutui a tasso agevolato per chi ha un'età compresa tra i diciotto e i con 5 dei 65 milioni di euro a disposizione destinati esclusivamente a coloro che avviano un'attività nel settore nei Comuni interessati dal sisma del 2016. Infine, come previsto dalla legge di bilancio, per gli *under* 40 che aprono un'azienda agricola è già prevista l'esenzione totale per tre anni dal versamento dei contributi previdenziali. Queste politiche danno il segno dell'importanza del ricambio generazionale nel settore agricolo, che significa non solo raccogliere il testimone dei genitori, ma anche e sempre più avvicinarsi alla vita agreste provenendo da altri settori o da diversi vissuti familiari e aspirando a diventare agricoltori di prima generazione. L'Unione europea, con la PAC e i Piani di sviluppo rurale, sostiene questi processi, creando opportunità di insediamento nell'agricoltura italiana per almeno 20.000 giovani fino al 2020. Si tratta di un grande progetto per dare nuovi stimoli al rinnovamento dell'agricoltura e alla competitività delle imprese.

La mozione a prima firma Formigoni catalizza positivamente l'attenzione del Governo sulle nuove sfide che la Politica agricola comune è chiamata ad affrontare nell'immediato futuro e sulle grandi direttrici di sviluppo e riforma degli anni a venire. Oggi siamo chiamati, come sistema Paese, a immaginare risposte di medio-lungo periodo su larga scala, ma anche a dare strumenti a favore del comparto agricolo, in modo che gli imprenditori agricoli possano trarre immediato vantaggio da tutte le opportunità garantite dalla PAC. L'Italia è da sempre protagonista del settore agricolo in Europa e nel mondo e deve essere in grado di far sentire la propria voce e porsi, ancor più nell'anno di presidenza del G7, come guida per una definitiva e duratura rinascita agricola.

Dico così perché ovviamente sappiamo che questo dibattito è già stato rinviato più volte, quasi che non fosse all'ordine del giorno l'importanza della nostra agricoltura

anziché partecipare all'assemblea annuale di Cisambiente era ad un incontro pubblico del suo partito, il Partito Democratico, proprio nel mio paese, a Tradate, negli stessi orari, negli stessi giorni e negli stessi momenti.

Ad esempio, c'è un'impostazione che vuole far passare i contributi, che oggi sono a fondo perduto, in strumenti finanziari. La nostra è un'agricoltura che non ha bisogno di sussidi, è un'agricoltura che non ha bisogno di sussidi, ma di sostegno; certamente non è un'agricoltura che si vuole e si deve sottomettere a delle valutazioni, a delle considerazioni a delle scelte finanziarie, altrimenti metteremmo un cappio al collo alle nostre piccole imprese che non hanno dimensioni strutturate per poter sostenere finanziamenti e soprattutto per poter contrarre rapporti con gli istituti di credito, come stabilito nella nuova PAC. A questo proposito, bisogna tenere conto anche delle difficili situazioni nelle quali opera la nostra agricoltura: spesso e volentieri è un'agricoltura pioniera, un'agricoltura che non abbandona il territorio, là dove fare agricoltura è praticamente antieconomico.

In questa relazione c'è una tabella riassuntiva molto efficace. Signor Presidente, in Francia c'è una superficie agricola di 27 in Italia ci sono circa 12 milioni di ettari. Ma è il numero di aziende che fa impressione, perché in Francia le aziende agricole sono 472.000, mentre in Italia si arriva al milione. Questo dà l'idea della differente struttura di un'azienda agricola e della differente relazione tra l'azienda agricola stessa e il territorio. È evidente che, in fase di modifica della PAC, il Governo si deve impegnare affinché gli elementi premianti tengano conto di queste differenze. Se invece la PAC viene costruita e modellata in funzione di strutture di agricoltura che non sono le nostre e che non tengono conto del grande valore aggiunto che l'agricoltura italiana dà a tutto il prodotto europeo,

Cito testualmente, sempre dalla stessa relazione. In Francia ci sono circa 27 milioni di ettari coltivati, mentre nel nostro Paese sono circa 12 milioni. 472.000 imprese, mentre dall'altra un milione. È evidente che questi numeri dicono che l'agricoltura italiana deve essere considerata per la sua peculiarità e non per la sua estensione. Spesso, signor Presidente,

che chiedeva all'Esecutivo di impegnarsi a modificare la nostra normativa, affinché il titolo di conduzione non sia più un limite alla percezione dei contributi europei. Purtroppo ancora oggi, su questo tema, ci troviamo ad aspettare un'azione da parte del Governo. Non lasciamo che la burocrazia soffochi la nostra agricoltura! riguardo alla Politica agricola comune e alla connessa mozione da noi presentata, va precisato che, sin dalla costituzione della Comunità economica europea, l'agricoltura ha rappresentato un settore economico avente valenza comunitaria. Non a caso, proprio la PAC è stata la prima e principale politica veramente comune sostenuta a livello europeo. Secondo la nostra visione, tuttavia, la PAC - nonostante le profonde trasformazioni subite negli anni - rimane afflitta da alcune criticità. In primo luogo, non è stato risolto il problema della squilibrata distribuzione degli aiuti. Prima della riforma del 1992, l'80 per cento del sostegno andava al 20 per cento degli agricoltori, mentre dopo il completamento di tale riforma (cioè nel 2005), cento degli agricoltori riceveva il 78 per cento degli aiuti. Più o meno immutate sono rimaste anche le contraddizioni legate all'eccessiva industrializzazione dei processi produttivi agricoli: le monocolture e gli allevamenti intensivi continuano ad essere diffusamente praticati e le misure agroambientali le misure agroambientali sono state utilizzate più dalle forme di agricoltura meno favorite rispetto a quelle ad alto grado di intensità che, come evidente, ne avrebbero avuto maggior bisogno. Tra le nuove criticità, va detto che il sistema di pagamento degli aiuti diretti al reddito, essendo stato concepito in relazione a dati storici relativi al possesso di fattori produttivi (cioè aiuti per ettaro o per capo di bestiame) ha favorito lo sviluppo di inevitabili fenomeni di rendita, che solo di recente iniziano ad essere considerati come da correggere. Il sistema a due pilastri, sebbene in misura minore, ha perpetrato lo storico squilibrio tra politica dei prezzi e politica delle strutture, tanto è vero che, ancora oggi, alle politiche di sviluppo rurale è riservato meno del 25 per cento delle risorse comunitarie, ossia meno del livello minimo che era stato indicato per gli interventi a sostegno delle strutture nella Conferenza di Stresa Il modello multifunzionale che l'attuale PAC dichiara di voler sostenere non si riferisce, in realtà, ad una agricoltura in grado di svolgere più funzioni oltre a quella produttiva. In questo si dimentica che il presidio ambientale è assicurato dalla presenza di attività agricole, che utilizzano in modo responsabile e sostenibile le risorse disponibili e non da forme improduttive, che si limitano a svolgere le pratiche necessarie per ricevere gli aiuti comunitari. L'attuale assetto della PAC, proprio perché determinato dalle spinte alla globalizzazione, non è più una politica che può essere considerata come la sintesi delle istanze provenienti dai Paesi membri. Ciò, tra le altre cose, pone importanti problemi riguardo alla democraticità dei processi decisionali che, di fatto, da tempo si sono spostati dalla sede comunitaria alle sedi internazionali, dove l'Unione europea negozia attraverso la Commissione, che tutto è fuorché una istituzione che risponde alle regole della rappresentanza democratica. La totale dipendenza della PAC alle regole del WTO - incluse quelle sulla proprietà intellettuale, che hanno determinato la formazione di oligopoli nel settore delle biotecnologie e, quindi, dei principali fattori produttivi agricoli posto seri problemi al mantenimento sul territorio sia delle attività agricole specializzate (che sono sempre più esposte alla concorrenza globale), sia dell'agricoltura delle aree interne cui, spesso, non resta altro che rinunciare a produrre e percepire gli aiuti comunitari concessi in base alla condizionalità. Bisogna inoltre avere presente che le attuali difficoltà economiche e sociali non sono le cause della crisi che stiamo vivendo, ma gli effetti dell'applicazione di un modello di sviluppo di tipo liberista e industrialista che, nel contesto della globalizzazione, ha potuto operare per circa venticinque anni, in modo assolutamente incontrollato (e quindi non governato) dalla politica. Per tali ragioni, è necessario che i futuri percorsi di crescita siano riferiti ad un modello alternativo a quello che ci ha condotto al disastro attuale e che, per quanto riguarda il ruolo dell'agricoltura, vi sia concretamente la possibilità che essa divenga il catalizzatore di modelli di sviluppo territoriale fondati sulla creazione di benessere diffuso (quindi il più possibile inclusivo), attraverso la valorizzazione delle risorse locali. Concludendo, solo in questo modo la PAC potrà costituire un concreto sostegno per il comparto primario e, nello stesso tempo, una parte davvero integrante della nostra politica

diversi interventi che colgono vari aspetti delle tante problematiche che la nostra agricoltura sta sopportando ormai da troppi anni. Debbo anche rilevare che se da un lato, in questa lista di *desiderata*, ci sono - come dicevo - molti dei punti che l'agricoltura vorrebbe vedere realizzati, è anche vero che poi ci deve essere la volontà da parte del Governo di trovare le forme corrette, efficaci e veloci per poterli realizzare, corriamo il rischio di parlare tra di noi, di parlarci addosso - come si suol dire - con un risultato pressoché inutile in questo confronto. anche questa volta debbo rilevare l'assenza del ministro Martina, senza nulla togliere alla figura del Vice Ministro, che forse ha la colpa, in senso positivo, di essere troppo presente,

agricola del nostro Paese. Probabilmente anche lui si fa condizionare da questa tendenza all'assenteismo che oggi si va manifestando; ma se nei cittadini può esservi una sorta di libertà di scelta, da parte del Ministro, invece, deve esserci un obbligo,

dire che gli agricoltori, i giovani e tutti coloro che stanno investendo non hanno bisogno di una burocrazia che li porti continuamente ad aspettare aiuti che non arrivano. Pertanto, cosa si chiede in questo bell'elenco di *desiderata*? di *desiderata*? Cosa chiediamo alla Politica agricola comune e al Ministro che non c'è (ma per fortuna c'è il Vice Ministro)? Chiediamo trasparenza nei mercati; chiediamo le stesse regole; chiediamo che venga valorizzato e garantito un prodotto; chiediamo dignità

quelle figure che invece dovremmo sempre ringraziare, perché non sono solo individui che fanno impresa, ma persone che preservano il nostro territorio e il nostro ambiente e che oggi si stanno impegnando per valorizzare il territorio e l'ambiente, anche attraverso l'agriturismo. Quindi, teniamo seriamente in considerazione, signor Vice Ministro sempre presente (a differenza del Ministro), che l'agricoltura ha bisogno di essere ascoltata, ha bisogno di tempi certi e non ha bisogno di burocrazia.

onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno attiene al futuro dell'Unione europea e, in particolare, a una delle politiche storiche su cui si è fondato il processo di integrazione europeo.

ed è in forse, per il periodo successivo, l'esistenza stessa di un Politica agricola comune, come dimostra il fatto che diversi Stati europei sono dell'idea di ridurre il *budget* stanziato per il settore agricolo, attualmente pari a circa il 38 per cento dell'intero bilancio della Comunità europea. Addirittura c'è chi propone di riportare la gestione dell'agricoltura a livello nazionale. Di per sé, la Commissione sembra intenzionata a proseguire nel percorso avviato sin dal 1962, tant'è che il presidente Juncker ha detto che le parole chiave del futuro in agricoltura sono «semplificazione» e «ammodernamento», mentre il commissario Hogan ha precisato che la PAC dovrà garantire alcune regole base per «assicurare una maggiore resilienza dei mercati, una produzione agricola più sostenibile e un migliore ricambio generazionale». D'altra parte, la PAC è stata una delle principali politiche del mercato comune europeo e ha permesso di conseguire l'indipendenza alimentare del nostro continente. Un traguardo che molto spesso si dà per scontato ma che, in realtà, così scontato non è. è. Peraltro, sebbene essa conti meno del 2 per cento del PIL e del 5 per cento dell'occupazione dell'intera Unione europea, va sottolineato che si tratta, in termini assoluti, di un settore che interessa circa 22 milioni di agricoltori e crea 44 milioni di posti di lavoro.

da una parte l'uscita del Regno Unito dall'Unione; dall'altra, le scelte di politica economica dell'amministrazione americana. Al momento, è verosimile che la PAC non subisca un drastico ridimensionamento, ma è realistico attendersi una diminuzione delle risorse assegnate e una conseguente riduzione rispetto al recente passato, degli obiettivi e degli strumenti. Qui entra in gioco l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Al di là del lungo percorso e delle ripercussioni che avrà sull'intero processo di integrazione europea, l'uscita del Regno Unito avrà certamente l'effetto di mutare gli equilibri del bilancio comunitario. Dall'altro lato e nel contempo, però, l'assenza del Regno Unito gioca a favore del mantenimento della Politica agricola comune, dal momento che i britannici prediligono un approccio marcatamente liberista e quindi contrario sia all'intervento di sostegno e di regolazione dei prezzi, sia alle politiche di tutela della qualità e dell'origine, viste da loro come un *vulnus* ai meccanismi del libero mercato. Potenzialmente determinanti per il futuro della Politica agricola comune saranno, poi, le scelte di politica economica assunte dall'amministrazione americana di Trump, che non ha mai fatto mistero delle sue idee protezionistiche. Un ritorno a politiche di stampo protezionistico non sarebbe sicuramente positivo per il nostro Paese, in ragione del ruolo che da sempre svolge il settore agroalimentare nel quadro della nostra bilancia commerciale. agricolo è stato determinante, tanto da fungere da traino negli anni della crisi, grazie al fatto che il settore ha dimostrato una forte competitività nei prodotti di alta qualità. Il protezionismo non sarebbe positivo neanche per i possibili effetti che avrebbe sul mercato interno. È vero che i dazi doganali rendono più costose le importazioni - a tutto vantaggio della produzione nostrana - ma sortiscono effetti analoghi anche per i nostri prodotti, la cui penetrazione nei mercati esteri sarebbe a questo punto ostacolata. Nel complesso, l'impressione generale è che da queste scelte la bilancia commerciale sarebbe fortemente penalizzata. In un siffatto contesto politico ed economico appare appare di tutta evidenza la necessità di intervenire sul settore agricolo con interventi ben mirati. La riforma della Politica agricola comune deve rispondere, oggi più che mai, alle nuove sfide che il recente panorama comunitario e internazionale ci chiamano ad affrontare. L'Unione europea, con misure che sappiano valorizzare la distintività territoriale delle produzioni, deve premiare l'occupazione delle aree rurali escludendo insostenibili rendite

Innanzitutto è necessario rafforzare tutte le misure che escludono la rendita dai benefici di Politica agricola comune, premiando di contro la capacità imprenditoriale e innovativa, al fine di ottenere alti *standard* qualitativi dei prodotti e delle aziende produttrici per riacquistare appetibilità sui mercati internazionali. Occorre poi implementare le produzioni di eccellenza agroalimentari nazionali sostenendo e tutelando la distintività dei prodotti *made in Italy*. Occorre creare un diffuso sistema di coordinamento di schemi specifici in ambito agro ambientale valorizzando così le peculiarità dei singoli territori e consentendo la cooperazione e l'aggregazione di imprese, per favorire l'accesso alle misure di sostegno a tutti gli operatori coinvolti, molti nel nostro Paese di piccole dimensioni. Infine, occorre promuovere il ricambio generazionale è una battaglia che stiamo sostenendo da tempo - mediante l'accesso a specifiche misure di sostegno all'imprenditoria innovativa condotta da giovani e dalle donne imprenditrici agricole.

per via di un macchinoso sistema burocratico e di restrittivi criteri selettivi. Spero che questa sia la direzione che riusciremo a seguire e a sostenere.